Comunico che in data 15 settembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dal Ministro dell'università e della ricerca* «Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» sospendo ora la seduta fino alle ore 18,30, per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia per il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, in corso di svolgimento presso la Camera dei deputati. È questo anche il motivo per cui

una nuova finestra"). Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 19 settembre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni Grazie a tutti Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi; nella Regione Basilicata: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Gianni Rosa e Mario Turco; nella Regione Calabria: Nicola Irto, Tilde Minasi, Mario Occhiuto, Fausto Orsomarso, Ernesto Rapani e Roberto Maria Ferdinando Scarpinato; nella Regione Campania: Vincenza Aloisio, Anna Bilotti, Susanna Lina Giulia Camusso, Gianluca Cantalamessa, Maria Domenica Castellone, Francesco Castiello, Giulia Cosenza, Raffaele De Rosa, Dario Franceschini, Antonio Iannone, Ada Lopreiato, Domenico Matera, Orfeo Mazzella, Luigi Nave, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Matteo Renzi e Francesco Silvestro; nella Regione Friuli-Venezia Giulia: Luca Ciriani, Marco Dreosto, Tatiana Rojc e Francesca Tubetti; nella Regione Lazio: Giulia Bongiorno, Nicola Calandrini, Peppe De Cristofaro, Cecilia D'Elia, Andrea De Priamo, Claudio Durigon, Claudio Fazzone, Maurizio Gasparri, Alessandra Maiorino, Lavinia Mennuni, Ester Mieli, Andrea Paganella, Raffaella Paita, Stefano Patuanelli, Cinzia Pellegrino, Marco Scurria, Filippo Sensi e Marco Silvestroni; nella Regione Liguria: Lorenzo Basso, Gianni Berrino, Roberto Menia, Luca Pirondini e Stefania Pucciarelli; nella Regione Lombardia: Alessandro Alfieri, Renato Ancorotti, Alberto Barachini, Alfredo Bazoli, Stefano Borghesi, Grazie Grazie a tutti Adriano Paroli, Daisy Pirovano, Isabella Rauti, Massimiliano Romeo, Licia Ronzulli, Elena Sironi, Sandro Sisler, Cristina Tajani, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata e Giusy Versace; nella Regione Marche: Guido Castelli, Roberto Cataldi, Antonio De Poli, Elena Leonardi e Alberto Losacco; nella Regione Molise: Costanzo Della Porta e Claudio Lotito; nella Regione Piemonte:

Grazie a tutti Valeria Valente e Ignazio Zullo; nella Regione Sardegna: Sabrina Licheri, Marco Meloni, Marcello Pera, Giovanni Satta e Antonella Zedda;

Antonino Germanà, Pietro Lorefice, Dafne Musolino, Nello Musumeci, Antonio Nicita, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvatore Sallemi e Daniela Ternullo; nella Regione Toscana: Claudio Borghi, Susanna Donatella Campione, Ilaria Cucchi, Silvio Franceschelli, Mariastella Gelmini,

Antonio Guidi, Walter Verini e Francesco Zaffini; nella Regione Valle d'Aosta: Nicoletta Spelgatti; nella Regione Veneto: Bartolomeo Amidei, Anna Maria Bernini, Mara Bizzotto, Luca De Carlo, Aurora Floridia, Matteo Gelmetti, Barbara Guidolin, Beatrice Lorenzin, Andrea Martella, Andrea Ostellari, Daniela Sbrollini, Raffaele Speranzon, Erika Stefani, Paolo Tosato, Adolfo Urso e Pierantonio Zanettin. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni. Su richiesta del relatore e secondo intese intercorse tra i Gruppi, la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge recanti iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, all'ordine del giorno della seduta di oggi, è rinviata alla prossima

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

del senatore Romeo, sulla promozione della pratica sportiva nelle scuole e sull'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, approvato dalla 7a Commissione lo scorso 3 agosto. Il provvedimento è frutto di un esame svolto in sede redigente e particolarmente approfondito, che ha consentito di arricchire il testo iniziale attraverso il contributo trasversale di tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione. Grazie anche all'accoglimento di numerosi emendamenti, è stato possibile pervenire ad una disciplina ampiamente condivisa, come testimonia il voto unanime, sul mandato a riferire favorevolmente oggi in Aula. L'articolo 1 stabilisce finalità ed obiettivi della proposta legislativa. Innanzitutto esso mira a promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico. La seconda finalità è il riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine si intende promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'attuazione di tali finalità è perseguita tramite la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù». L'articolo 2 istituisce i citati i giochi, la cui promozione e organizzazione è curata dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene al riguardo prevista la possibilità, da parte del Ministero, di avvalersi della società Sport e Salute Spa, sentite le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP). Possono partecipare ai giochi tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie, in modo che sia favorita un'equa rappresentanza di genere; l'unico vincolo è che siano regolarmente iscritti e frequentanti. In sede di esame in Commissione è venuta infatti meno la previsione che limitava la partecipazione ai giochi agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che avessero ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva stessa. La definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei giochi e per la relativa partecipazione degli studenti è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con le autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità. A seguito delle modifiche introdotte in Commissione, per gli studenti con disabilità è ora prevista la partecipazione sia a gare integrate, sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione. Inoltre il decreto ministeriale istituisce una sezione dedicata a sport di squadra, dove studenti con disabilità e normodotati possano giocare insieme. Ai sensi dell'articolo 3, lo svolgimento dei giochi è coordinato a livello nazionale... Grazie, Presidente. Ai sensi dell'articolo 3, lo svolgimento dei giochi è coordinato a livello nazionale dalla Commissione organizzatrice nazionale. Essa è composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità Alla Commissione spettano la redazione dei regolamenti annuali per lo svolgimento dei giochi e l'individuazione delle sedi, d'intesa con le commissioni organizzatrici regionali. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale, nonché la sua articolazione articolazione a livello regionale, sono definiti da un successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza delle scuole primarie, con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e una seconda a livello provinciale, riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. Nel corso dell'esame in Commissione, oltre a essere stata introdotta la fase d'istituto, è venuto meno il carattere agonistico della fase provinciale. La seconda sezione in cui si articolano i giochi è denominata «Nuovi giochi della gioventù» ed è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado. Tale sezione si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolata nelle sessioni estive e invernali. La disciplina dell'attività sportiva per la partecipazione ai giochi è contenuta nell'articolo 4: nello specifico, si stabilisce che gli istituti scolastici si possano collegare in rete con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti per la stipula di protocolli annuali e pluriennali con gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento delle delle discipline sportive. Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività sportive dovranno essere volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti scolastici della scuola secondaria, le attività sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive in quanto occasione da utilizzare in un momento sportivo come competizione tra gli alunni e l'agonismo è inteso come impegno a dare il meglio di sé e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive. Ai suddetti protocolli è demandata l'individuazione, tra l'altro, delle modalità di svolgimento dei corsi, delle sedi di svolgimento delle attività sportive, delle tappe di percorso formativo e dei criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi, dei criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi, delle modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi e delle eventuali forme di sponsorizzazione da parte di imprese, ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti senza scopo di lucro. Nel corso dell'esame è stato espunto il riferimento ad eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva. L'articolo 5, introdotto in Commissione, reca disposizioni in materia di prevenzione sanitaria. Nello specifico, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche, delle associazioni tecnico-scientifiche e delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani che partecipano ai Giochi della gioventù. Infine, l'articolo 6 dispone l'avvio in forma sperimentale dei giochi per l'anno scolastico 2024-2025 ed individua la copertura degli oneri finanziari derivati da tale provvedimento. Signor Presidente, Ringrazio il presidente Romeo per essere stato il primo firmatario di questa importante proposta, ringrazio tutti i Gruppi che sono stati presenti in Commissione - quindi in Parlamento - per aver contribuito in maniera importante

Grazie a tutti i colleghi

Signor Presidente, colleghi, membri del Governo,

devo dire una cosa. Oggi, in maniera straordinaria, il dottor Croce e i suoi collaboratori hanno contribuito a ridurre il numero delle barriere architettoniche in questo Senato un po' ostile alle persone con difficoltà motoria e sensoriale. È un grande successo. Non è un favore a me, ci mancherebbe, ma è il Senato che sta cambiando, anche a livello di fruibilità, di accessibilità e, se vogliamo, di rispetto degli altri, da qualsiasi punto di vista si possa leggere. *(Brusio).* anche quella di far comprendere le idee partitiche diverse. È un esempio di "tolleranza", che dovrebbe servire anche a noi, ad essere più accessibili ad accettare l'idea degli altri, senza affatto rinunciare ai propri contenuti partitici e politici.

se qualcuno mi conosce, sa che parlo talmente tanto che la fatica non c'è. È che faccio fatica a farmi comprendere. credo che la forma peggiore di dissenso sia quello del brusìo disconfermante. Entro velocemente

la Commissione di merito, il presidente Marti, il presentatore del disegno di legge, ma anche i tre Ministri coinvolti, in particolare per quanto mi riguarda

Poche volte, signor Presidente, ho visto una collaborazione così efficace, in cui anche le distanze partitiche hanno fatto un passo indietro per portare avanti questo provvedimento. Signor Presidente, colleghi, lo sport, soprattutto nelle scuole,

facevano ginnastica, attività fisico-motoria e sport, mentre io ero confinato, quasi carcerato, in aula a disegnare brutte cose col gesso alla lavagna, quasi per sentirmi occupato. Quel dolore lo porto ancora e stasera veramente penso di avere - permettetemi di dirlo

nell'antica Grecia e persino in momenti oscurissimi dell'ultimo periodo bellico; soprattutto, però, per quello che ci riguarda, non conosce razzismi, non conosce l'utilizzo infame delle cosiddette diversità: nello sport, per fortuna soprattutto in quello minorile e adolescenziale, si è tutti uguali applauditi nel vincere, ma anche quando si perde se c'è buona volontà. Avviandomi alla conclusione con un po' di rammarico, perché questo è un argomento che mi affascina molto, sia per il vissuto personale che per la mia attività di neuropsichiatra, credo che oggi segniamo una grande vittoria, perché anche in un momento difficile a livello economico e - se vogliamo - anche a livello sociale e culturale, merito soprattutto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche nostro in tutte le configurazioni, noi dimostriamo che, nonostante le difficoltà contingenti anche economiche, si può guardare, si può concretizzare la speranza dell'oggi e del domani. Questa pure è un'attività sportiva dal punto di vista politico politico e partitico. Un ultimo punto per me è fondamentale. Il presidente Marti ha usato più volte, come sempre ottimamente, la parola «disabilità» valorizzandone il diritto-dovere alla partecipazione. Questo è un argomento fondamentale, perché dà il segno che nello sport non ci sono differenze etniche, culturali, religiose, né diversità legate al proprio stato psicofisico. *(Applausi)*. Ho visto, e concludo, persone sordo-cieche nuotare e appassionarsi per vincere: è una dimostrazione di coraggio e, se ce ne fosse bisogno, avremo modo tutti noi

con serenità e, se possibile, guardando un po' avanti, cosa che non sempre viene fatta. Viva la vita, vita lo sport.

non si mette in discussione il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie per questo provvedimento, in particolare non il mio, visto che ero presente a una finale nazionale dei Giochi della gioventù nell'età in cui avevo

non ci si esime dall'usare quel linguaggio permeato di leggera ipocrisia che è tipico della scuola quando parla di sport. Lo sport è agonismo e sana competizione, mentre da sempre la scuola cerca di far passare la componente educativa, che ovviamente è l'obiettivo della scuola, come preponderante rispetto all'agonismo. Insomma, la competizione non piace tanto agli insegnanti e questo traspare da questo testo faccio un esempio: all'articolo 1, comma 2, si parla di confronto culturale e sportivo. Mi perdoni, signora Presidente, ma il confronto sportivo è è sempre culturale, anzi, è la cultura - come diceva il senatore Guidi - del partire tutti dalla stessa linea di partenza e dall'essere tutti uguali. Lo sport è cultura in sé, non c'è lo sport e la cultura.

Al mondo di oggi c'è l'abitudine più che a fare ad apparire e qui mi sembra che sia appaia due volte, mentre si fa una volta sola e anche questo probabilmente merita una riflessione. All'articolo 5 poi, come ha ha illustrato il relatore, viene istituito un tavolo di lavoro cui partecipano rappresentanti delle società sportive più rappresentative, delle società scientifiche, delle associazioni tecnico-scientifiche e delle professioni sanitarie, che sono tutti più o meno enti privati.

non è previsto neanche un rimborso spese. Allora, come al solito nel nostro Paese, si cerca di fare le nozze con i fichi secchi: non si può pensare che della gente venga a Roma a partecipare a una commissione *gratis* e pagandosi la benzina.

di questo argomento, che molti di noi considerano davvero importante, alla presenza di giovani studenti. Quando il lavoro su un testo legislativo viene portato a compimento con il voto unanime della Commissione di riferimento, possiamo dire di aver scritto davvero una bella pagina della nostra politica. Seppure con i distinguo necessari che appartengono alla dialettica parlamentare e al confronto - e ben venga - questo però è quanto è accaduto in 7a Commissione cultura e sport proprio in merito a un disegno di legge come quello allora, prima di tutto, di ringraziare il presidente Marti, tutta la Commissione, la nostra vice presidente Giusy Versace e tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito al testo. Parliamo di una legge di tutti proprio perché, durante i lavori della Commissione, sono stati accolti emendamenti proposti dai partiti anche dell'opposizione, inclusi i nostri e non era affatto

non solo un sano stile di vita, ma anche un prezioso strumento educativo oltre che di inclusione sociale. Anche per questo siamo felici del fatto che ci sia stata la volontà di ripristinare i Giochi della gioventù, scelta che certo non basta rispetto alle tante cose utili che dovremmo fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Occorre certamente più aiuto alle scuole; bisogna stanziare più fondi se si vuole davvero promuovere la pratica sportiva e creare nuove opportunità di crescita per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. Del resto, i primi Giochi della gioventù, nati nel 1969 per volontà di Giulio Onesti, che allora era Presidente del CONI, avevano proprio questo obiettivo. Allo stesso tempo, dovevano servire per sensibilizzare le nuove generazioni su altri aspetti importanti della loro vita, quali appunto una sana alimentazione, stili di vita corretti, il rispetto dell'ambiente, delle regole e per la persona e favorire l'inclusione sociale. Sono tutti temi questi di cui anche oggi continuiamo a parlare e di cui abbiamo un disperato bisogno, anche in virtù dell'aumento di quella difficoltà e di quel disagio giovanile che abbiamo visto esplodere ancora di più dopo gli anni della pandemia. Serve quindi un lavoro legislativo corale. Negli anni, i Giochi della gioventù hanno consentito a milioni di studenti di praticare uno sport gratuitamente, educandoli e favorendo la pratica di svariate discipline, e sono stati molto spesso una vera e propria palestra, fucina che ha partorito campioni, medaglie olimpiche e paraolimpiche, di cui l'Italia anche oggi deve essere fiera. Eppure, una manifestazione così importante, incardinata nelle tradizioni scolastiche dell'Italia, è stata sospesa già due volte nel corso della storia recente, prima nel 1996, per poi essere ripresa nel 2007, e poi fermata definitivamente nel 2017 a causa di una costante riduzione del numero dei partecipanti, appena 400.000. È evidente che occorre chiedersi dove si è sbagliato: il taglio dei fondi, la formazione dei docenti, la mancanza di collaborazione tra scuola ed enti di promozione?

di intervenire sulle croniche criticità esistenti che non sono poche - penso alle infrastrutture scolastiche, spesso piene di barriere architettoniche - che poi non sono in grado ovviamente di mettere in moto la macchina organizzativa. A mio avviso, però, questa sarà la sfida più difficile, considerando la mancanza di palestre e di aree dedicate allo sport e se consideriamo, come molti di noi che hanno presentato anche testi di legge, lo sport, l'attività fisica come un potente farmaco naturale che non ha controindicazioni, un farmaco che fa bene a tutte le età e che va prescritto in ricetta medica. Dobbiamo evitare allora che si creino scuole di serie B e scuole di serie A, soprattutto se si pensa che le infrastrutture - come prevede il testo - dovranno accogliere anche gli studenti con disabilità. Dobbiamo allora lavorare tutti insieme uniti per abbattere ogni forma di barriera ed evitare che si realizzi uno scenario di questo tipo. tipo. Pur non facendo parte della 7a Commissione, come responsabile sport di Italia Viva so quanto importante sia questo aspetto. allora lavorare affinché i nuovi Giochi della gioventù vedano la luce nell'anno scolastico 2024-2025; motivo per cui viene istituita una commissione per l'organizzazione composta dal Dipartimento dello sport, dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dal Ministero dello sport e della salute, dal CONI e dal CIP. dunque un grande e serio gioco di squadra per superare le tante criticità e le tante barriere che ancora permangono da Nord, Centro, Sud. Prima di concludere, colgo l'occasione per ricordare che finalmente domani, alla Camera dei deputati, in ultima lettura si voterà la riforma costituzionale che prevede l'inserimento della pratica sportiva all'interno della nostra Carta costituzionale. Credo che anche questo vada veramente applaudito come un segnale di unità del Parlamento: un passaggio epocale, quanto mai necessario, proprio a voler sottolineare che anche il diritto allo sport viene riconosciuto, tutelato e garantito dalla nostra Repubblica; un diritto, così come il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, all'interno dell'articolo 33 della Costituzione, e quindi all'interno del diritto all'istruzione, con l'aggiunta di un nuovo comma. Allora, per festeggiare domani, con l'auspicio di avere alla Camera i numeri necessari per arrivare a questo importante risultato, auspichiamo tutti assieme di scrivere un'altra pagina importante, oggi e domani, anche per una seria e giusta riforma

il disegno di legge in esame è molto importante - a mio avviso - perché pone la pratica sportiva al centro del processo di formazione degli studenti nelle scuole. L'educazione sportiva nelle scuole nella storia, anche in quella delle civiltà antiche, ha rivestito un ruolo significativo nella formazione dei cittadini, e non solo per la salute e il benessere, ma anche in generale, in stretta connessione con la filosofia. Entrambe infatti, filosofia ed educazione allo sport, cercano di sviluppare l'individuo in modo completo, combinando aspetti fisici, mentali e spirituali. La filosofia greca antica enfatizzava il concetto di eudemonia, il raggiungimento della felicità e del benessere attraverso la virtù e l'ottimizzazione delle potenzialità umane. I Giochi olimpici antichi erano visti proprio come un mezzo, attraverso la competizione leale, per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza fisica e mentale. Gli antichi romani avevano un'enfasi sulle virtù militari come la forza, la disciplina e il coraggio, e insegnavano questo attraverso l'addestramento fisico. Il taoismo, una filosofia cinese antica, promuove l'armonia con il *tao*, che è il cammino, attraverso l'equilibrio e l'azione spontanea. Il Tai Chi - vediamo spesso anche qui in Italia dei cinesi che lo praticano nelle piazze - è una forma di ginnastica cinese che si basa su questi principi. Il confucianesimo enfatizza l'importanza della moralità, dell'etica e del comportamento corretto: principi applicati nello sport attraverso la promozione del *fair play*, del rispetto per gli avversari e della disciplina personale, come sa bene il mio collega Lotito. Durante il periodo dei samurai, il *bushido* era il codice etico seguito dai guerrieri giapponesi che includeva virtù come l'onore, il coraggio e la disciplina. Nei monasteri Shaolin dei monaci buddisti, ancora oggi le arti marziali sono considerate una via per comprendere i principi come la compassione, la non violenza e la ricerca dell'illuminazione, sviluppando in armonia mente e corpo. In quasi tutte le civiltà l'educazione sportiva era uno dei pilastri fondamentali di una connotazione culturale con profonde radici culturali, sociali e spirituali. Queste tradizioni sportive hanno contribuito a definire le identità e i valori delle comunità nel corso della storia, ma non è un fatto scontato. In Italia oggi si assiste, al contrario, a una diminuzione della pratica sportiva nelle scuole da parte dei giovani. A volte, persino l'ora di ginnastica viene saltata e utilizzata per altri scopi. Ci sono dei motivi culturali: l'Italia ha una lunga tradizione accademica e culturale, la quale però potrebbe aver messo in secondo piano l'importanza dello sport come parte integrante dell'educazione. Inoltre, assistiamo alla sempre maggiore diffusione di olimpiadi di giochi elettronici, così come a pericolose *performance* su TikTok; diminuisce, di contro, quell'immagine del ragazzo che alla sera, dopo gli studi, torna a casa con il suo zaino pieno di indumenti sudati. Ci sono anche dei motivi strutturali: il sistema scolastico italiano è carente delle risorse necessarie, e una tale carenza di finanziamenti e di strutture, che esiste soprattutto nel Mezzogiorno, può ostacolare l'implementazione di programmi sportivi nelle scuole. Non si parte da zero - è vero - ma c'è molto da fare, se consideriamo che quattro complessi scolastici ogni dieci non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva. Con il PNRR sono stati destinati circa 300 milioni di euro agli impianti sportivi, di fronte però a una richiesta da parte dei Comuni di circa 3 miliardi; quindi saranno necessarie ulteriori risorse. In Europa ci sono invece Paesi in cui la pratica sportiva nelle scuole è massimamente promossa e incentivata: in Finlandia e Svezia, ad esempio, gli studenti partecipano a lezioni di educazione fisica quasi tutti i giorni. Anche in America tutti conoscono il ruolo significativo che le università americane hanno nello sport e gli atleti possono ottenere borse di studio per competere nei migliori *college*. Si capisce facilmente allora perché investire in programmi sportivi nelle scuole è un investimento nel benessere e nella formazione dei futuri cittadini. Promuovere lo sport nell'ambito della scuola e in quell'età dove la coscienza è ancora predisposta a immagazzinare valori sani come la cura della propria salute, la leale competizione, la solidarietà verso il compagno di squadra, è una scelta di campo con smisurati e potenziali effetti benefici e fa il paio con quella che amiamo definire costituzionalizzazione dello sport, che è già *in itinere*, come ricordava la collega Sbrollini. È uno strumento eccezionale per affrontare le disabilità motorie, ma anche per infondere quella forza psicologica a coloro che sono rimasti vittime di incidenti. La previsione di uno specifico percorso di competizione sportiva a valenza nazionale nell'ambito del cammino scolastico porterà a un ulteriore impulso anche verso una coscienza diffusa sul ruolo che lo sport ha nella cura della salute, concorrente in modo vitale al benessere fisico e psicofisico. Lo scopo dei Nuovi giochi della gioventù è di essere il più possibile inclusivi. Viene creato un collegamento tra la scuola e l'attività sportiva, anche al di fuori delle ore tradizionali di lezione. È quella che chiamiamo la scuola al centro del villaggio: non solo una scuola con attività formative, ma anche una scuola che si apre alla comunità e ai soggetti più svantaggiati, soprattutto nei quartieri degradati. A tal fine viene proposta la collaborazione fra le istituzioni scolastiche e i Nuovi giochi, che vengono istituiti per consentire ai ragazzi di partecipare alle varie discipline sportive. Proprio partecipare ci sembra il termine chiave: ai Nuovi giochi della gioventù possono partecipare tutti. L'altra implicazione immediata è quella sulla salute dei più giovani, come dicevo prima. Attivare la più ampia partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività sportive significa spesso toglierli dalla sedentarietà. Promuovere uno stile di vita attivo può certamente avere implicazioni positive sulla loro salute e sul fatto di evitare ovvero affrontare meglio in futuro alcune patologie. anche fare in modo che diventino degli adulti più sani. Insomma, la partecipazione allo sport dei più giovani è anche un investimento sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario nei prossimi anni, posto che la maggior parte delle patologie possono essere evitate o controllate con successo. Un ragazzo su quattro risulta essere sovrappeso, anche a causa di un'attività sedentaria passata spesso davanti ai dispositivi elettronici tipo *videogame* o telefonini. Quella della maggiore divulgazione dello sport tra i giovani è pertanto una vera e propria sfida per il futuro, utile per prevenire malattie croniche e migliorare la salute negli ultimi vent'anni di vita, stimolando le persone verso percorsi di invecchiamento attivo sin dall'adolescenza. Il disegno di legge di cui oggi discutiamo, pertanto, è il segno tangibile dell'attenzione di questa maggioranza. Per questo ringrazio anche il presidente Romeo, la Commissione e tutti quelli che hanno lavorato, il presidente Marti i Ministri. È importante e necessario creare una rete sempre più diffusa di soggetti capaci di preparare un futuro di benessere e salute fisica e mentale, iniziando dalle politiche attive nelle scuole, che sono il primo contesto dove la persona si affaccia, uscendo dal guscio della propria famiglia, e poi si forma. È quindi un disegno di legge che quindi noi valutiamo con estremo favore e al quale va il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

intervenga nelle sedi internazionali - in queste ore i nostri rappresentanti, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri sono all'ONU - sul problema del Nagorno-Karabakh. È una grande questione umanitaria, e è una grande questione politica. L'Azerbaigian ha rotto gli indugi nei confronti di una popolazione stremata,

*(Applausi)*. Noi chiediamo che le Nazioni Unite facciano sentire la loro voce e si avvii un'azione multilaterale per far sedere a un tavolo Armenia, Azerbaigian e tutti i grandi *player* dell'area, dalla Turchia alla Russia, all'Unione europea, che purtroppo non vediamo proprio così presente come vorremmo. Tutti debbono in qualche modo facilitare una soluzione, che non può essere un'*escalation* militare. Non vorrei che, con il fatto dell'Ucraina e dell'incredibile conflitto a cui stiamo assistendo, ci fosse una sorta di parallelismo acquiescente che consenta di fare azioni inaccettabili nei confronti del popolo armeno. Il popolo armeno non ha risorse straordinarie dal punto di vista del gas o di altri altri prodotti naturali di questo tipo, che hanno una grandissima importanza nella geopolitica. Ma l'Armenia ha una grande storia e una grande tradizione e il suo popolo ha già subito nella sua storia pagine terribili di genocidio. Noi vorremmo che il Governo italiano faccia sentire la propria voce e anche il Parlamento, tramite la Commissione esteri, voglia esprimere una

Chi conosce la storia delle vicende in questione sa che il *Nagorno-Karabakh* vive una guerra civile strisciante dalla fine degli anni Ottanta. come fu simbolico per tutta Europa il 1989, la caduta del muro di Berlino e la caduta del comunismo. Dalle rovine dell'Unione sovietica nacque pure questa vicenda. Il *Nagorno-Karabakh* è notoriamente abitato nella quasi integrità da popolazione di origine armena, tant'è che dalla dissoluzione dell'Unione sovietica alla formazione dei diversi Stati, quella che prima era la comunità di Stati indipendenti, il *Nagorno-Karabakh* chiese di essere annesso a quella che era la Repubblica ex socialista sovietica di Armenia. L'Armenia nel frattempo è diventata un'altra cosa: grazie a Dio non solo la Repubblica socialista di allora, ma ha rivendicato orgogliosamente i suoi natali. L'Armenia è il primo Stato cristiano d'Europa, prima di Roma, novant'anni prima di Teodosio. L'Armenia per chi la visita è un territorio straordinario, con i monasteri incastonati nella roccia, e il *Nagorno-Karabakh* è la stessa cosa. Chi ascolta una messa armena pensa di pensa di essere in pieno Medioevo cristiano o di ascoltare il gregoriano, ma questo evidentemente non basta. Da quella che era una guerra civile strisciante siamo arrivati a una situazione che si è evoluta fino a ciò che sta accadendo oggi.

La gente sta morendo, i bambini muoiono, le medicine e i generi alimentari non ci sono. Noi ovviamente ci preoccupiamo Ci sono sempre Paesi più importanti che non i deboli. Quando venivano sterminati dai turchi degli armeni non si accorgeva nessuno e non piangeva nessuno e sta accadendo anche adesso, nel silenzio dell'Europa e del mondo. Quello che sta accadendo nel *Nagorno-Karabakh* è semplicemente indecente e antiumano. Ecco perché mi associo alle parole del presidente Casini e dico qualcosa di più.

e le cose vanno dette chiaramente. Si sa chi è colpevole e chi è colpito. Da una parte c'è una grande Nazione, che tra l'altro è molto ricca, perché ha gas, ha petrolio ed è islamica; dall'altra parte c'è una piccola Nazione che ha testimoniato la cristianità in Europa e nel mondo e ha sofferto purghe spaventose, verso la quale abbiamo il dovere e il diritto di manifestare la nostra solidarietà. *(Applausi)*. Lo faccia il Parlamento, facciamolo tutti insieme e lo faccia il Governo italiano. Cerchiamo di essere protagonisti in quella che deve diventare evidente - una questione di carattere internazionale che coinvolge tutto il mondo civile e il mondo che crede a questi valori. Signor Presidente, io intervengo per fatto personale, a fine seduta, come prevede il Regolamento. Mi riferisco alla seduta di giovedì scorso, durante il *question time*, quando il ministro Tajani, rispondendo a una interrogazione, che non era quella che gli avevo rivolto io, ma quella successiva, le seguenti parole, che sono a verbale della seduta: «Mi spiace che il senatore Scalfarotto, che è così interessato ai problemi della Libia, quando si parla di un disastro abbia abbandonato l'Aula; forse ci seguirà attraverso la televisione, com'è suo costume». Quindi, il Ministro degli affari esteri dice in quest'Aula che il mio costume è seguire le sedute in diretta televisiva, da casa. Ora, posto che

non è il Governo che controlla il Parlamento e le presenze dei parlamentari; è il Governo che, quando viene qui, si sottopone al controllo del Parlamento. Il rapporto fiduciario intercorre tra il Parlamento e il Governo e, quando il Governo viene in quest'Aula, è pregato di rispondere alle interrogazioni con puntualità, cosa che il Ministro non ha fatto. La stizza di questa sua reazione, di questo fallo a gamba tesa, dimostra la posizione di qualcuno che non era stato in grado di rispondere all'interrogazione precedente.

dalla Presidenza di turno che, quando un episodio di tal genere accade, sia la Presidenza a tutelare l'onorabilità del Parlamento e a spiegare al Ministro che questo tipo di uscite non gli sia consentito; quando viene in quest'Aula, grazie alla fiducia della quale egli è Ministro, dovrebbe avere il rispetto che si deve ai rappresentanti del popolo che qui siedono: cosa che lui non ha fatto. che comprendo la stizza e il dispetto di essere stato messo in difficoltà da un'interrogazione alla quale non ha saputo rispondere. Capisco che il Ministro è portatore di una politica estera molto debole, molto debole, che sta mettendo in difficoltà questo Paese. Questo atteggiamento, però, non gli deve essere consentito. Io la pregherei, per il futuro, di adoperarsi, anche personalmente, insieme ai suoi colleghi Vice Presidenti e al presidente La Russa, per spiegare qual è il rapporto che intercorre tra il Parlamento e il Governo, che è un rapporto di controllo. Eravamo in sede di di sindacato ispettivo. Era il Parlamento che rivolgeva una domanda al Governo e il Governo non può, per il rispetto che deve a quest'Aula, permettersi uscite come quella che il ministro Tajani

di magnitudo 4.9, con epicentro nel comune di Marradi; un sisma avvertito, molto forte, anche nei comuni vicini, quali Tredozio, Modigliana, Portico, San Benedetto, Brisighella; un sisma che, fortunatamente, ha fatto non vittime, ma solo lievi danni, come crolli di cornicioni, lesioni ad alcuni edifici, sia pubblici che privati, che naturalmente poi si è provveduto a fare evacuare per sicurezza; un sisma, però, che è avvenuto negli stessi territori in cui si è abbattuta l'alluvione pochi mesi fa, su una popolazione già fortemente provata. Ecco perché ho chiesto di intervenire oggi, a fine seduta, per esprimere vicinanza e solidarietà a queste popolazioni, a nome non solo mio, ma anche di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, con l'augurio che lo sciame sismico si sia risolto nella giornata di ieri e i nostri concittadini possano così tornare a dormire tranquilli in casa propria e nei propri letti. *(Applausi)*.